con comunicazione del 18 settembre, il senatore Vincenzo Cuomo ha dichiarato di optare per la carica di sindaco della città di Portici. Trattandosi di un caso di opzione derivante da una situazione d'incompatibilità, il Senato ne prende atto. Autorizzo la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a convocarsi per procedere all'accertamento relativo all'individuazione del candidato subentrante.

PLI))*. Signor Presidente, arriviamo alla discussione di queste mozioni purtroppo con qualche ritardo oggettivo rispetto ai lavori

per introdurre alcune delle misure al centro della discussione che svolgeremo di qui a breve in quest'Assemblea sul tema sia dell'allargamento sul tema sia dell'allargamento della platea dei rimborsi agli obbligazionisti sia delle sanzioni rispetto ai comportamenti tenuti dagli amministratori che si sono resi responsabili del fallimento di alcune banche nel recente passato.

e, quel che è peggio, al Senato, essendo sopraggiunta la necessità per il Governo di chiedere la fiducia sul provvedimento, non è stato più possibile cambiare il testo che ci era

per fare un buon lavoro, emendando il lavoro fatto dal Governo con un atto d'indirizzo, invitando il Governo stesso al primo provvedimento utile, la prossima legge finanziaria, a sanare alcune questioni che sono state al centro del dibattito e delle aspettative della pubblica opinione nei mesi delle polemiche roventi sul destino dei risparmiatori travolti dal *crack* delle banche.

norme che dovrebbero consentire al giudice di applicare sempre la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti di questi signori.

le loro considerazioni sulla progressione che ha portato all'esclusione ingiusta di questi obbligazionisti e ad un trattamento fin troppo morbido nei confronti dei responsabili dei fallimenti. Emerge qui una questione politica,

una catena di avvenimenti che ha lambito persino la credibilità stessa del Governo (non è mia abitudine accentuare gli aspetti che determinano *pruderie* che coinvolgono parenti e conoscenti di membri del Governo, su cui non voglio quindi quindi soffermarmi), c'è una grande distanza tra il modo in cui alla fine si è deciso di affrontare la situazione e ciò che era giusto e lecito concedere alle aspettative di centinaia e migliaia di risparmiatori increduli e della più vasta opinione pubblica, a cui sostanzialmente è stato spiegato che non si poteva andare oltre

Sono state due non risposte inspiegabili e non spiegate di fatto dal Governo, su cui oggi è necessario tornare. Tornandoci, il Senato compie esattamente il suo dovere, dovere, con un atto di indirizzo che corregge ed emenda queste lacune nella condotta del Governo di fronte all'emergenza che ha colpito il Paese e migliaia di famiglie. Purtroppo, registriamo con qualche amarezza la presentazione di un altro documento da parte della maggioranza - in particolare del Partito Democratico - in cui, ancora una volta, queste due questioni vengono totalmente eluse

nel fallimento e nella rovina una parte non trascurabile del nostro sistema bancario. Questi sono i due cardini della partita che si svolgerà in quest'Assemblea nelle prossime ore e credo che, a fronte di questa situazione, non possiamo che ribadire il nostro massimo impegno in Assemblea per arrivare a concludere quel risultato che è stato troppo a lungo negato sia all'opinione pubblica, sia ai risparmiatori.

ordine di Banca Intesa Sanpaolo a cui il Partito Democratico, il Governo e la maggioranza politica hanno ritenuto di voler soggiacere, con buona pace delle prerogative del Parlamento. In Commissione finanze alla Camera dei deputati, tuttavia, il relatore, ovvero un membro di questa maggioranza, aveva presentato un emendamento, aveva presentato un emendamento, che poi è stato ritirato forse perché ci si è resi conto che riguardava tutti gli amministratori delle banche fallite, quindi compresi anche gli amministratori di Banca Etruria, particolarmente protetti dal Partito Democratico. Tale emendamento intendeva, in primo luogo, ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari del fondo di solidarietà in secondo luogo, prevedeva norme volte a irrogare adeguate sanzioni per consentire al giudice di condannare gli amministratori delle banche, banche, qualora ritenuti responsabili, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il ritiro dell'emendamento da parte del relatore e la successiva fiducia non hanno consentito il dibattito su questi temi nelle Aule parlamentari. Questa condotta ha leso gravemente le prerogative del Parlamento, che si è trovato, quindi, depotenziato e privato della sua funzione primaria.

a favorire il più ampio dibattito - diversamente da quanto è stato fatto finora - su questi temi, anche al fine di definire una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite;

banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

salva banche si è affermato come interesse primario solo ed unicamente la stabilità del sistema bancario rispetto ai creditori sociali e questo è il principio che sovrintende all'azione del Governo ed anche - devo dire - all'azione di Bankitalia e della Consob, per i quali la tutela dei risparmiatori è l'ultimo dei pensieri.

amministratori, ampliava i criteri per il rimborso agli obbligazionisti subordinati delle banche venete. È quindi un tema sul quale vi è molta attenzione, perché ovviamente c'è la questione non risolta del ristorno verso i risparmiatori

Vorrei ricordare che recentemente c'è stato un pronunciamento da parte della Corte di cassazione che ancora una volta assolve, ad esempio

invece, come ho già detto, con la scusa della fiducia ha voluto evitare questo tema, evidentemente anche per grandi imbarazzi politici. Speriamo che con queste mozioni e con gli impegni che queste indicano al Governo oggi l'Assemblea del Senato possa fare un passo in avanti.

e dare un senso compiuto a quello che stiamo facendo, occorra ancora soffermarsi sulle ragioni di tali atti di indirizzo.

recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca, si aprì un dibattito attorno a due questioni fondamentali: il primo riguardava una sorta di *par condicio* risarcitoria

forte di giustizia nei confronti di quegli amministratori che si fossero resi colpevoli di azioni contrarie alla buona gestione. In quella discussione e nel passaggio in Commissione, il relatore presentò un emendamento che non venne posto in votazione immediatamente e che riproduceva integralmente

affermava che, ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La *ratio*, l'obiettivo di questo emendamento era che, di fronte a un'accertata responsabilità degli amministratori delle banche oggetto di dissesto, agli stessi fosse sostanzialmente impedito di reiterare condotte analoghe di elevato disvalore sociale. Il citato emendamento ebbe sostanziale parere positivo del Governo; nel passaggio in Assemblea, come è stato ricordato, l'Esecutivo scelse un'altra strada, cioè quella di presentare nel maxiemendamento il testo originale senza alcuna correzione.

finanze del Senato del 18 luglio scorso in un'audizione del ministro Padoan sulle questioni bancarie, di fronte a un'osservazione e a una domanda specifica del nostro capogruppo Cecilia Guerra,

a carico degli operatori del settore bancario, considerata l'esigenza di evitare e quindi eventualmente di reprimere il verificarsi di condotte scorrette».

alla Camera e sia conseguente alle dichiarazioni che il ministro Padoan ha reso in Commissione finanze al Senato. Credo che ci sia lo spazio per trovare - questo è un nostro auspicio una sintesi unitaria e più ampia possibile perché su questo tema - concludo, riservandomi di intervenire in dichiarazione di voto - occorre avere la consapevolezza che siamo di fronte - molti colleghi oggi presenti

tra i consumatori, i risparmiatori, il sistema bancario e le istituzioni. È una ferita talmente profonda - lo voglio dire con grande che non si può pensare di curare con pannicelli caldi, e cioè con espressioni che rimandino a un tempo indefinito l'applicazione delle pene accessorie, che rischiano rischiano di essere controproducenti e, anzi, di essere vissute come una sorta di presa in giro. C'è, in altri termini, una domanda di giustizia - è il senso della nostra

l'economia e i sistemi bancari sa che la fiducia è un capitale immateriale, spesso però più importante dei parametri economici e degli indicatori imposti dagli organi di vigilanza. Ciò che ci aspettiamo è una posizione del Governo che apra sul tema e sia coerente - come dicevo con le dichiarazioni rilasciate prima dell'estate, perché dobbiamo provare a sanare la ferita. Questo sarebbe un primo passo nella direzione della giustizia.

onorevoli colleghi, sottosegretario Baretta, le ragioni della discussione di questa mattina sono state ampiamente ricordate dai colleghi. Solo per continuità voglio ricordare che con il citato decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito in legge nel mese di luglio, è stato compiuto un ulteriore e decisivo passo verso la completa stabilizzazione del nostro sistema bancario e che tale intervento fa seguito alle misure adottate per la risoluzione di quattro banche e la ricapitalizzazione preventiva del Monte dei Paschi di Siena. Siamo qui a discutere di una questione, come ricordavano i colleghi, legata alla perseguibilità degli amministratori, alla ricerca anche di un equilibrio risarcitorio, che rimane un tema, a mio parere, necessario. Voglio solo ricordare, prima di arrivare ai punti salienti che ci hanno indotto a presentare come maggioranza questa mozione, che è in corso un'ampia disamina delle proposte di modifica delle disposizioni relative alla gestione delle crisi bancarie in ambito europeo relativa, in particolar modo, alla direttiva sulle risoluzioni degli enti creditizi e su quella sui requisiti patrimoniali. Ciò avviene 6a Commissione permanente del Senato sta partecipando con la definizione sia di risoluzioni sia di atti in fase ascendente, sulle quali la Commissione stessa, come ricorderanno i colleghi che ne fanno parte, ha ipotizzato un pronunciamento dell'Assemblea proprio per andare incontro alle esigenze ricordate. Inoltre, ricordo che, anche in base alle risultanze delle indagini conoscitive condotte dalla Commissione finanze del Senato, la gestione del credito, anche nelle banche venete, presentava irregolarità e e scarsa valutazione del rischio di credito; che lo *status* di banca popolare, nello specifico, era stato utilizzato per adottare comportamenti che andavano nel senso della scarsa trasparenza e della irresponsabilità

che i tentativi del *management* di tenere a galla la banca aveva dato vita a pesanti pressioni su correntisti e affidatari per l'acquisizione di azioni per valori che sono poi crollati in pochi mesi. mesi. Parte di questa discussione, ovviamente, potrà essere sviluppata nella Commissione di inchiesta sul sistema bancario italiano. Atteso, però, che, a normativa vigente, esiste un problema di percezione nell'opinione pubblica di sostanziale mancanza di incisività in termini di sanzioni dei comportamenti irregolari, illeciti o fraudolenti degli amministratori e che, nonostante le misure di ristoro anche nei confronti dei detentori di obbligazioni lo ricordo - sono strumenti finanziari diversi dalle azioni, ma comunque con carattere di investimento di rischio e ben diversi dai depositi), resta l'esigenza di ricostruire un saldo rapporto di fiducia con le banche e anche, come ha ricordato chi mi ha preceduto, un saldo rapporto che sani quell'ampia quell'ampia ferita con alcuni territori del nostro Paese che è sotto gli occhi di tutti. Per questo abbiamo predisposto un atto che impegna il Governo su cinque punti: a favorire in tempi rapidi una ricognizione del complesso delle norme sanzionatorie, sia di rango penale che di al fine di verificarne l'adeguatezza, tenendo conto del quadro normativo dell'Unione europea in materia, compresa, per quanto riguarda le banche beneficiarie di aiuti di Stato, la *banking* *communication* del 2013; a verificare l'opportunità di introdurre misure finalizzate a collegare, nei casi di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori all'irrogazione di sanzioni nei loro confronti per condotte illecite e fraudolente; ad assumere iniziative, con il coinvolgimento delle autorità nazionali di vigilanza, per garantire la corretta applicazione, da parte di tutti i soggetti abilitati a prestare servizi di investimento, delle regole finalizzate ad impedire il collocamento degli strumenti finanziari più rischiosi presso clienti al dettaglio non in grado di comprenderne l'effettivo rischio, e al contempo a rafforzare le sanzioni per il mancato rispetto di tali regole; ad avviare iniziative per la promozione e l'effettiva diffusione dell'educazione finanziaria; infine, a istituire, in accordo con le istituzioni dell'Unione europea e nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un veicolo speciale per assistere le banche nell'opera di pulizia pulizia dei bilanci, in grado di creare un mercato dei crediti deteriorati, il cui smobilizzo ordinato, nel medio periodo, costituisce la strada maestra per restituire risorse all'economia reale e ridare capacità di credito alle banche.

che adesso non vediamo più), si diceva che le banche erano una casta ed erano usurai. Cosa significa questo? Che c'era una ristretta oligarchia che gestiva le banche, che ovviamente favoriva i propri amici e gli amici degli amici e che tartassava il risparmiatore

alla Camera dei deputati aveva proposto un emendamento sulla base del quale si sarebbe disciplinato un inasprimento

oltre che l'ampliamento della platea degli obbligazionisti cui estendere i benefici previsti dal fondo di solidarietà, rimodulando il termine di acquisto dei titoli dal 12 giugno 2014

chi erano i cento più importanti debitori che hanno fatto saltare le banche, perché, conoscendo quelli, si può fare la diagnosi. Sono un medico e

fallite o in fallimento (perché ce ne sono tante altre); a fare tutto quanto nelle proprie possibilità per garantire i risparmiatori degli istituti bancari falliti dopo il 1° febbraio 2016 (e non già dopo il il 12 giugno 2014), al pari di quanto quindi previsto per i beneficiari del decreto-legge possibile per i risparmiatori la partecipazione ai processi di liquidazione degli istituti di credito in fallimento. Crediamo che se arrivassero queste risposte

il rapporto delle banche con i propri clienti e la funzione che il sistema bancario svolge in un Paese democratico e soprattutto in appoggio all'economia. Credo infatti che il Parlamento e il Governo debbano sciogliere un equivoco di fondo riguardo alle trasmissioni televisive sulle banche. Ve ne sono infatti in cui le banche vengono accusate di non assumersi rischi per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia

conto del fatto che prima poi la crisi finirà e che c'è chi, anche onestamente e con tutte le buone intenzioni del mondo, pensava di poter investire e continuare a produrre, ma si è trovato in una situazione nella quale la crisi è continuata per anni. Vi poi altre trasmissioni televisive, in cui viene sostenuta la tesi assolutamente contraria e cioè che gli amministratori, nel momento in cui il credito che è stato erogato non può essere recuperato, sono oggettivamente responsabili di quello che è accaduto e devono essere quindi chiamati a rispondere alla sbarra, anche personalmente, penalmente e civilmente, dei danni che hanno provocato. Credo allora che il Parlamento e il Governo debbano chiarire, nella vicenda che ha coinvolto tante banche italiane, due situazioni totalmente diverse. Da una parte ci sono gli amministratori delle banche che hanno avuto dei problemi, dall'altra gli amministratori delle banche che non solo hanno avuto problemi, ma che hanno tenuto comportamenti illeciti o che comunque hanno sostenuto iniziative fuori dalla realtà, in cui evidentemente c'erano dolo, malafede e la consapevolezza che il credito erogato non avrebbe fatto ritorno, o che hanno venduto agli ignari clienti

fare attenzione a non criminalizzare un intero sistema e a non coinvolgere anche gli amministratori per bene, che hanno sostenuto una linea

Presidente, non ho ben chiaro su cosa indagherà. Forse si costituirà e passerà le carte alla prossima legislatura. Credo dunque che ci debba essere anche la volontà di arrivare a fare questi chiarimenti, di arrivare a fare questi chiarimenti, senza guardare in faccia a nessuno e, quindi, andando davvero a verificare le responsabilità, anche penali, dei singoli, ma facendolo con un minimo di concordia all'interno dell'Assemblea e con tempi che consentano un risultato utile soprattutto ai risparmiatori, ovvero a coloro che hanno innocentemente subìto questa situazione e che chiedono una risposta positiva dalle istituzioni.

Gli interventi di stabilizzazione del sistema bancario, che, con diverse modalità, hanno affrontato le diverse situazioni di crisi del nostro sistema creditizio, hanno certamente avuto come obiettivo primario quello di introdurre criteri più stringenti e rigorosi di gestione, al fine di evitare, per quanto possibile, il manifestarsi di futuri elementi di criticità. Come sappiamo, vi sono tre principali problemi. Il primo è costituito dal peso crescente sui bilanci bancari dei crediti deteriorati, il secondo problema è individuabile in un deterioramento della redditività e, per finire, c'è una sempre più rilevante esigenza di ricapitalizzazione. Ciò ha reso necessari interventi che fossero in grado di assicurare adeguati livelli di liquidità, il ripristino della capacità di finanziamento e, inoltre, la definizione delle necessarie misure di rafforzamento patrimoniale delle banche. È stato certamente importante prevedere la possibilità di concedere la garanzia dello Stato in ordine alle passività degli istituti di credito italiani. È un'assunzione di forte responsabilità, che ha in parte restituito fiducia ai mercati di fronte ad una condizione di sofferenza strutturale, che sarebbe stata ancor più grave se esposta ad una ulteriore svalutazione dei crediti in sofferenza. Al tempo stesso si è operato affinché il livello degli accantonamenti e delle garanzie reali, in rapporto alle sofferenze lorde di cui parlavamo in precedenza, fosse adeguato. In ambito europeo la riflessione è certamente aperta, in primo luogo per quanto attiene alla trasparenza dei bilanci degli istituti di credito e all'esigenza di favorire un sistema bancario solido. Le politiche poste in essere per incidere positivamente sulle crisi bancarie sono state adottate in coerenza con le modalità di intervento rese possibili dagli indirizzi e dalle disposizioni dell'Unione europea, in particolare con riguardo proprio all'esigenza di porre in essere interventi risolutivi delle crisi senza ricorso a risorse pubbliche. Si è operato quindi, con tali vincoli, attraverso il Fondo interbancario, a garanzia prioritaria dei depositi e, dunque, dei correntisti. È evidente che in Italia sia particolarmente acuta l'esigenza di riformare il sistema sanzionatorio in presenza di comportamenti illeciti e irregolari da parte di coloro che amministrano gli istituti di credito e sia indispensabile rafforzare il nostro sistema di vigilanza. È un fattore decisivo per restituire fiducia ai risparmiatori, che di certo è stata pesantemente intaccata dalla collocazione sistematica di strumenti finanziari ad elevato rischio, se non di titoli allocati in modo fraudolento da parte di istituti di credito in dissesto, da irregolarità e comportamenti irresponsabili adottati in violazione delle regole proprie di un mercato ordinato e trasparente.

sostenere la ricerca di risorse private, i cui esiti dipendono dalla risposta dei mercati e dall'evoluzione dell'economia reale; occorre quindi liberare, almeno in parte, le banche sane dagli oneri di mutualità imposti dagli istituti in crisi; infine evitare la formazione di ulteriori perdite che determinerebbero una maggiore e sistematica sottrazione di risorse. gli indirizzi che nella fase immediata e, ancor più, nel medio periodo devono avere attuazione. Per concludere, condividiamo sia l'urgenza dei provvedimenti adottati a tale scopo, sia la considerazione che tale percorso sia necessariamente graduale ai fini della stabilità generale del sistema bancario. È quindi evidente che ciò debba avvenire con la consapevolezza che tale intervento debba essere strutturale e andare in profondità per dare finalmente stabilità ad un settore strategico per il rilancio della nostra economia e nella massima tutela di tutti i risparmiatori. Signora Presidente, la materia bancaria attraversa i nostri lavori come un fiume carsico, che appare e scompare. Decreti legge, interventi, tamponamenti, stanziamenti e, adesso, anche questa giusta richiesta - che ho sottoscritto,

Quando si sono fatti i vari provvedimenti e decreti, ogni volta si è rinviata ad altra fase l'azione punitiva e più decisamente sanzionatoria.

e poi ovviamente chi li presta ad altri deve farlo con le garanzie dovute. Tutto ciò non è avvenuto: si potrebbe parlare ore - ma qui non abbiamo il tempo per farlo - raccontando varie cose; ricordo che nella precedente legislatura il presidente *pro tempore* dell'ABI,

c'è stata un'assoluta non considerazione di un emendamento importantissimo,

composti principalmente da crediti verso le banche (3,8 miliardi), crediti in *bonis* verso la clientela (30,1 miliardi), attività finanziaria (8,8 miliardi) e per la parte restante di varia natura. Il gruppo creditizio guidato dall'amministratore delegato Carlo Messina ha altresì acquisito passività per complessivi 51,3 miliardi composti da debiti verso le banche (9,3 miliardi) e verso la clientela (25,8 miliardi) e titoli in circolazione 11,8 miliardi. Lo sbilancio tra attività e passività acquisite rappresenta un credito di Intesa nei confronti delle liquidazioni ed è stato provvisoriamente quantificato in 5,4 miliardi di euro. Questo si aggiunge a quello che era già accaduto per Banca Etruria e CariChieti. È evidente che stiamo operando che riguardano altro, altrimenti non ci saremmo trovati qui oggi a dover discutere mozioni che vanno a sanare quella che era una priorità non riconosciuta

un servizio alla popolazione. In Italia non solo non garantiamo la distinzione tra banche commerciali e banche che fanno interventi finanziari, ma continuiamo a tutelare chi sbaglia. Quello che, allora, andava fatto prioritariamente, cari colleghi, era proprio la ricognizione di tutta la normativa sanzionatoria

che non sia collegato alle banche, che abbia le mani libere e che sia in grado di riportare nella giusta misura e nella corretta dimensione la funzione e il ruolo delle banche cosicché i cittadini

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le mozioni oggi all'esame vengono discusse in un momento particolare, in cui molti fatti sono già accaduti, a fronte della grande vulnerabilità del sistema finanziario nazionale ed europeo, come effetto della lunga crisi iniziata nel 2007. Oltre al recentissimo decreto-legge che riguardava le banche venete, ci sono stati nei mesi scorsi passaggi significativi che hanno riguardato l'azione dell'Unione europea, che ha approvato molti interventi volti a definire una disciplina più rigorosa per quanto concerne i requisiti patrimoniali richiesti alle banche in modo da garantirne la solvibilità e ha gradualmente costruito l'architettura dell'unione bancaria, realizzando un sistema unico di vigilanza. Questo nuovo sistema, seppure con alcuni aspetti problematici relativi alla compressione degli spazi delle autorità nazionali, ha consentito l'armonizzazione dei criteri precedentemente rimessi alle singole autorità nazionali. Per quanto riguarda, poi, la risoluzione delle crisi bancarie, è stata definita una disciplina che possa contrastare gli effetti distorsivi legati a massicci salvataggi a carico dei bilanci pubblici con diversi strumenti. molte delle quali ad oggi in fase di attuazione, stanno contribuendo a rafforzare il sistema bancario nazionale - mi riferisco ai vari provvedimenti - benché l'elevata consistenza dei crediti in sofferenza e le ricadute delle normative europee sopra richiamate in tema di risoluzione rendano necessario accrescere la capacità di tenuta del sistema. dalla fine del 2015 l'Italia ha sperimentato, in accordo con le autorità europee, tre opzioni di intervento in materia bancaria: il cosiddetto *burden sharing*, con risoluzione, vendita delle banche risolte e rimborso nella forma più ampia permessa dei detentori di titoli subordinati, applicato nei casi di Banca Marche, la CariFerrara, la Banca Etruria e CariChieti; la ricapitalizzazione precauzionale con continuità aziendale e significativo ristoro dei detentori dei titoli come nel caso del Monte dei Paschi di Siena; la liquidazione amministrativa coatta con scorporo delle sofferenze e cessione ad un soggetto terzo, con risorse pubbliche e ristoro in forma analoga alle precedenti, applicato nei casi delle due banche venete. In relazione agli interventi sopra descritti è emersa una problematica non secondaria, che ha messo in evidenza comportamenti gravi e poco trasparenti e una tendenza marcata al rischio eccessivo da parte degli amministratori delle suddette banche che in molti casi ha avuto come vittime, purtroppo, la clientela *retail*, i piccoli correntisti e gli azionisti delle medesime banche. Temi, questi, che saranno al centro dei lavori della Commissione di inchiesta in via di insediamento. Numerosi sono i casi di strumenti finanziari collocati dalle banche in violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione da parte di soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario nelle due banche. Nel caso delle banche venete in particolare, i risparmiatori clienti delle banche si sono ritrovati, loro malgrado, azionisti delle banche o possessori di titoli obbligazionari. In molti casi le banche hanno condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei clienti - mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cosiddetti mutui soci, riservati appunto ai soci - all'acquisto di proprie azioni od obbligazioni convertibili, soprattutto nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale negli anni 2013 e 2014. La prassi seguita da queste banche aveva l'obiettivo di collocare titoli presso i richiedenti credito per conseguire l'aumento di capitale necessario a rispettare determinati coefficienti patrimoniali. patrimoniali. In sostanza, si riscontrano comportamenti assolutamente poco trasparenti degli amministratori, grande carenza di vigilanza il fatto che questo sia avvenuto richiama un cambiamento di normativa. Per questo la mozione fissa alcuni passaggi che riteniamo fondamentali: in primo luogo, come già detto, occorre effettuare, in tempi rapidissimi, una ricognizione del complesso delle norme sanzionatone, sia di rango penale che amministrativo, previste nel nostro ordinamento per i casi sopra menzionati per poterne verificare l'adeguatezza, tenendo conto anche del nuovo quadro normativo in sede europea. In secondo luogo, dopo questa ricognizione,

l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori all'irrogazione di sanzioni nei loro confronti per condotte illecite e fraudolente. In questo caso, è importante anche agire con quel sistema che nella legge fallimentare si chiama di revocatoria, con grande attenzione a misure dilatorie messe in atto da alcuni amministratori; si citava il caso, molto frequente, di chi ha separato i propri patrimoni dalla responsabilità nell'imminenza dell'irrogazione delle sanzioni:

ad impedire in futuro il collocamento degli strumenti finanziari più rischiosi presso clienti al dettaglio non in grado di comprenderne l'effettivo rischio. Un secondo passaggio fondamentale è quello di agire, in accordo con le istituzioni dell'Unione europea e nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per trovare una soluzione al problema centrale che ferma lo sviluppo e il normale funzionamento del nostro sistema creditizio: i crediti deteriorati. In tale ambito, riteniamo indispensabile che venga istituito un veicolo speciale per assistere le banche nell'opera di pulizia dei bilanci, in grado di creare un mercato dei crediti deteriorati il cui smobilizzo ordinato, ordinato, nel medio periodo, costituisce la strada maestra per restituire risorse all'economia reale e ridare capacità di credito alle banche. Infine, non è secondario il tema richiamato nella nostra mozione, quello della promozione e della diffusione dell'educazione finanziaria tra i cittadini, in quanto le vicende che abbiamo visto hanno coinvolto numerosi risparmiatori, con ingenti perdite di capitale investito, evidenziando in molti casi, oltre alle gravi carenze degli amministratori e della vigilanza, una impreparazione di fondo nei confronti dei prodotti finanziari acquistati e la mancanza

Signor Presidente, le mozioni presentate sostanzialmente affrontano due problemi: la responsabilità degli amministratori e la tutela dei risparmiatori. Francamente, sulla responsabilità degli amministratori

il senatore Fornaro nel suo intervento ha giustamente detto che la forza di una mozione su questo punto è direttamente proporzionale all'ampiezza del consenso del Senato. Vi è un secondo punto, più delicato, che concerne la tutela del risparmiatori, perché impatta molto con le regole europee, con il quadro di riferimento europeo. Su questo tema, anch'esso presente in tutte le mozioni,

noi. L'auspicio è che la Conferenza dei Capigruppo possa valutare una definizione sufficientemente rapida della conclusione della discussione, anche alla luce del tentativo che il sottosegretario Baretta si impegna a promuovere. Questa decisione però competerà

problema è la tempistica, nel senso che non ci sfugge, dalla memoria recente, un lungo trascinamento di queste mozioni nelle settimane e poi nei mesi d'attesa. Per noi va benissimo attendere attendere questa proposta, che valuteremo con attenzione e con rigore, perché comunque per noi ci sono due punti fermi non superabili, non nella forma ma nella sostanza, il il problema è che effettivamente si giunga poi a una votazione in un tempo molto ravvicinato, ragionevolissimo: tra una settimana al massimo. Dobbiamo concludere questa vicenda, anche perché l'ultimo tram che passa

aderiamo a questa impostazione senza dimenticare, però, che abbiamo grandi perplessità sulla volontà del Governo di arrivare a una soluzione. Nessuno di noi può dimenticare che sul provvedimento delle banche venete alla Camera dei deputati in Commissione VI il relatore, in accordo con il Governo, aveva presentato un emendamento

che le nostre mozioni diventino fatti concreti risiede nell'eventualità che alle prossime elezioni la maggioranza cambi e ci sia qualcuno meno disponibile a mettere un pietoso velo

abbiamo soltanto la legge di bilancio in cui riuscire a inserire degli emendamenti e delle norme. Spero quindi che tutti i Capigruppo concorderanno che c'è l'urgenza di approvare queste mozioni e di inserirle

Signor Presidente, anche noi aderiamo alla proposta del sottosegretario Baretta, che condividiamo nel merito e anche nel giusto proposito di cercare una condivisione massima sul tema, visto che partiamo da un insieme di mozioni che pongono in modo analogo, se non talvolta addirittura uguale, questi aspetti molto problematici e di grande interesse per l'intero Paese. Mi associo, però, alla volontà, che è stata già espressa, di chiarire che ci deve essere già in questa Aula un impegno di tutti i Gruppi a far sì che si arrivi a una conclusione della vicenda. Quindi, signor Presidente,

la necessità di verificare gli opportuni inserimenti, essendo stato corale l'invito in tale direzione ma dovendo compiere noi i passaggi procedurali Quindi, il Governo agisca indipendentemente dalla fissazione in calendario, che anche io mi auguro possa essere rapida, perché gli elementi sono stati tutti chiariti e messi sul tappeto dalla discussione.